L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in ordine all'affare inerente la revisione delle leggi elettorali. Ricordo che su tale richiesta può prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti. Seguirà poi la votazione per alzata di mano.

sono d'accordo con questa deliberazione. Il nostro Gruppo, coerentemente con il comportamento che ha sempre avuto per quanto riguarda l'impostazione

la necessità di affrontare la crisi della rappresentanza che oggi è un nodo fondamentale della crisi della politica. Abbiamo presentato, da più legislature, non solo in questa, disegni di legge che danno una precisa interpretazione della crisi della democrazia parlamentare che, a nostro giudizio, proviene da quell'errata impostazione, in un contesto quale quello del 1992, che fu l'introduzione del sistema maggioritario. Con il sistema maggioritario, in un passaggio a nostro avviso non rispondente all'impianto costituzionale, si è passati da una democrazia parlamentare, che quindi riconosceva al Parlamento la centralità il ruolo d'impulso (di formazione, per altro, del Governo), ad una democrazia governante in qualche modo basata un ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri molto presidenzialista, un ruolo in cui il Parlamento era ridotto a un insieme e, spesso, a un coacervo di interessi localistici. Il non completamento, peraltro, della riforma ci ha lasciato a metà del guado. Oggi ci troviamo a subire tutte le conseguenze negative di un'introduzione parziale di un sistema maggioritario, avendo perso avendo perso le caratteristiche che derivano, a nostro avviso, dallo stesso impianto costituzionale del sistema proporzionale. A questo punto, crediamo che bisogna discutere in Parlamento. Quando dico "in Parlamento" intendo dire che, trattandosi di regole del gioco istituzionali, bisogna confrontarsi tra maggioranza e opposizione e possibilmente giungere ad una normazione e, quindi, anche ad una nuova legge elettorale che veda la stragrande maggioranza dell'Aula d'accordo.

più o meno occulte di ostruzionismo che tendano, in qualche modo, a far svolgere il *referendum*, vanificando il ruolo del Parlamento

fortemente il ruolo della maggioranza e lo stesso Governo. Anche dal punto di vista tecnico della formazione della rappresentanza, una legge che scaturisse da un simil*e referendum*, ammesso che superasse i requisiti di costituzionalità - il che mi sembra molto incerto -, sarebbe alla fine una legge autoritaria e non risolverebbe nessuno dei problemi

trattativa che danno comunque un'utilità marginale e un valore di contrattazione ai singoli parlamentari e ai singoli Gruppi (spesso i più piccoli)

può pensare, colleghe e colleghi, che per facilitare la costruzione del Partito democratico si debba, con un corto circuito, semplificare la complessità del quadro politico in maniera autoritaria nei confronti non soltanto di piccole forze alleate, che pure vanno tutelate, ma anche di forze intermedie

una formula per farci tornare ad un sistema che, in qualche modo, coniughi ed interconnetta una formazione proporzionale democratica della rappresentanza - e ve ne é bisogno per ricostruire il ruolo centrale e prioritario del Parlamento con un'azione efficace di Governo. Vi sono dei sistemi che, in maniera anche comparata a livello europeo e non solo, potremmo studiare in 1a Commissione. Noi siamo per un sistema tedesco, riscritto ovviamente in forma italiana per le necessarie variazioni. Credo che sia possibile tenere insieme queste due identità di fondo: rappresentanza proporzionale di una società complessa, e quindi rappresentanza veritiera di questa società, e azione efficace di Governo. I due aspetti possono stare insieme e non si escludono a vicenda, come affermano

col contributo non soltanto della vecchia maggioranza, ma anche con il fondamentale contribuito della minoranza di allora, l'attuale maggioranza.

La più grande debolezza di questa legge è che di fatto ha nominato il Parlamento e ciò non accade nelle democrazie, ma nelle oligarchie:

che anche quando era in vigore la legge precedente si sapeva prima, collegio per collegio, chi sarebbe stato eletto da una parte o dall'altra.

probabilmente crea maggioranze diverse nelle due Camere. La maggioranza di allora presentò la legge con un sistema di calcolo da collegio unico nazionale anche al Senato, che poi fu costretta a correggere sulle pressioni di alcuni costituzionalisti che al Presidente della Repubblica facevano presente che non sarebbe stata una cosa corretta, dal punto di vista costituzionale. Eppure oggi sappiamo tutti che altri costituzionalisti sostengono esattamente il contrario, anzi nella mia proposta di legge - non quella di allora che immetteva semplicemente le preferenze alla legge vigente, ma quella più complessa che ho presentato all'inizio della legislatura prevede il premio di maggioranza al Senato con collegio nazionale e redistribuzione regionale, come vuole la Costituzione. Allora, la legge è una porcata per il contributo di maggioranza e minoranza; quindi, non mi alzerei tanto facilmente con questa critica, ma facciamo un'autocritica generale, mi ci metto anch'io, anche se fui l'unico insieme con il mio Gruppo a presentare le modifiche che avrebbero consentito già a quella legge di impedire la nomina dei parlamentari.

che in Europa non c'è legge che preveda un premio di maggioranza e qualcuno dei miei colleghi sottolinea

non fanno caso al fatto che in Europa non c'e legge che preveda insieme il premio di maggioranza e lo sbarramento. Quella sì che sarebbe una legge truffa: sbarramento e premio di maggioranza insieme sono un enorme premio di maggioranza che fa fuori 12 milioni di elettori italiani che si riferiscono ai loro partiti, cioè alle loro culture, i cosiddetti piccoli partiti, che con uno sbarramento al 4 per cento regalano rappresentanza per il 25 per cento del Parlamento a partiti che non vorrebbero votare.

E lo riconoscono tutti gli statisti europei. Perché non mettiamo intanto chiarezza sul minimo delle regole? Si può stare dalla parte di chi vuole il premio di maggioranza maggioranza e dalla parte di chi vuole lo sbarramento, ma non si può stare dalla parte di chi vuole lo sbarramento e il premio di maggioranza, perché o è ignorante colui che sostiene questa tesi, oppure è in malafede.

però i piccoli partiti rischiano, per difendersi dai grandi partiti che ragionano come ho detto poco fa, di finire sul *referendum*, che è una cosa oggettivamente vergognosa dal punto di vista democratico, perché il *referendum* è quello che vediamo oggi in Parlamento.

Questo vuole il *referendum* così modernista, così liberale, così innovatore? Ho l'impressione che i costituzionalisti che stanno dietro questo *referendum* non sappiano molto di Costituzione; purtroppo la situazione è minata all'origine, perché si vogliono i cartelli elettorali e più che mai oggi il centro-sinistra sa che questo non può più chiederlo né volerlo, perché insieme non ci possono stare. Allora, bisogna andare oltre. Bisogna pervenire ad una legge che non consenta semplicemente di stare insieme per avere

ai partiti grandi - perché è evidente che se i piccoli dovessero sospettare che saranno loro l'agnello sacrificale con i loro 12 milioni di cittadini italiani che li votano,

innanzi tutto i nostri apprezzamenti per gli sforzi compiuti sia dal Governo, in particolar modo dal ministro Chiti, che dall'opposizione, nella persona del senatore Calderoli, per riformare urgentemente il sistema elettorale in vigore. Autonomie ha partecipato ad ambedue le consultazioni, quella del Governo e quella del tavolo dei volenterosi convocato dal senatore Calderoli. Abbiamo anche presentato propri disegni di legge che perseguono l'obiettivo di eliminare le distorsioni evidenti, nonché - questo è il punto principale sul quale chiedo attenzione - riavvicinare l'elettorato agli eletti. L'obiettivo principale, infatti, che ha animato la discussione del nostro che reputo condivisibile da tutti - è quello di riportare la politica nel suo insieme ad un legame più stretto con la popolazione e con l'elettorato, che sempre più palesemente evidenzaun forte distacco da tutta la politica, non solo da quella della maggioranza, anche da quella dell'opposizione. Uno dei motivi principali che ha causato tale distacco risiede nell'attuale legge elettorale. Sono stati, infatti, aboliti i collegi uninominali che garantivano un diretto collegamento tra i candidati eletti nei collegi e gli stessi elettori. Si è tornati al proporzionale nella convinzione che esso che esso potesse garantire maggiori vantaggi in termini di rappresentatività e che potesse rispecchiare meglio i reali rapporti tra i vari partiti e le forze politiche. Purtroppo nulla di ciò si è verificato, anzi, al contrario, la legge ha prodotto un gravissimo distacco tra cittadini elettori, da una parte, ed eletti, dall'altra, tra corpo elettorale e rappresentanti in Parlamento ed ha, inoltre, reso maggiormente instabile il Governo, avendo riportato una esile maggioranza al Senato. La più grave limitazione del diritto dell'elettore è stata quella - sottolineo quanto detto dal senatore Cutrufo poco fa - di toglierli la possibilità di esprimere le preferenze. La normativa attualmente in vigore prevede liste bloccate dei candidati di ogni partito e, così facendo, ha tolto la possibilità ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, chiamandoli solo ad approvare elenchi decisi dai partiti.

La seconda forte critica riguarda le candidature plurime, ossia la possibilità data al candidato di presentarsi in più di una circoscrizione per poi optare per una di esse. Il cosiddetto eletto plurimo è signore del destino di tutti gli altri candidati la cui elezione dipende dalla sua opzione. Questo fenomeno coinvolge un terzo dei parlamentari. Il problema istituzionale causato dalla legge elettorale (oltre queste lacune) è la ulteriore frammentazione delle forze politiche e una situazione di non governabilità del Paese. Il Gruppo Per le Autonomie, nel raffronto dei vari sistemi elettorali di cui si è occupato in varie sedute e grazie alle esperienze degli anni passati, ha deciso di proporre in questa sede il sistema uninominale, prevedendo, per la Camera dei deputati, un sistema uninominale secco a turno unico, dividendo il territorio nazionale in tanti collegi quanti sono i deputati da eleggere.

due delle tre legislature elette con il sistema maggioritario, la XIII e la XIV, sono giunte alla loro scadenza naturale. Un ulteriore vantaggio è dato da un diretto legame tra l'eletto e l'elettorato. I piccoli collegi garantiscono conoscenza diretta dei candidati e la disponibilità degli stessi verso le istanze locali e le preoccupazioni della gente, superando proprio quel distacco e quel divario che si lamenta oggi nella politica. Il Gruppo Per le Autonomie si augura, pertanto, un sistema più vicino alla gente, un legame più diretto tra eletti ed elettori con un sistema maggioritario in collegi, se non esclusivamente almeno maggiormente uninominale.

a rispettare i princìpi fondamentali democratici della scelta dei candidati e della vicinanza tra candidati ed elettori. Se, pertanto, la maggioranza del Parlamento - e non parlo di maggioranza politica - dovesse decidere di conservare il sistema proporzionale con premio di maggioranza,

Ringrazio in questa sede sia il Governo che il senatore Calderoli per l'attenzione che ha dimostrato anche per le istanze delle minoranze linguistiche. È chiaro che l'applicazione di soglie elettorali senza distinzione verrebbe a ledere l'articolo 6 della Costituzione, che prevede espressamente la tutela delle minoranze linguistiche, ma su questo aspetto sono state date da tutti rassicurazioni. Riguardo poi al quesito dell'abbreviazione della procedura e dell'applicazione della procedura d'urgenza, intendo invece sottolineare che capisco e condivido pienamente l'urgenza di legiferare in materia elettorale, anche per prevenire il *referendum*. Non nascondo, una certa perplessità per quanto riguarda la riduzione dei tempi. Non vorrei che ciò si traducesse in una rinuncia ad un vero dibattito e ad un approfondimento, di cui una legge di tale importanza ha assolutamente bisogno.

il Parlamento abbia sia in sede di Commissione che in Aula il tempo necessario per approfondire la materia proprio al fine di scegliere la soluzione migliore per il Paese. La procedura d'urgenza dovrebbe pertanto essere intesa, secondo quanto richiesto dal senatore Calderoli,

ha anche bisogno di riforme costituzionali. Ho parlato della riduzione dei costi della politica; aggiungo di dare il diritto elettorale ai diciottenni anche qui al Senato al fine di equiparare il corpo elettorale. Si propone pertanto l'equiparazione del diritto di voto

di più. La diversità rispetto al maggioritario di collegio, che pure produce un effetto maggioritario, è che quando si vota in un collegio si pesa ugualmente sul voto finale. Si vince o si perde il collegio, e l'effetto maggioritario viene dal numero dei collegi che si sono vinti o si sono persi.

il premio di maggioranza fa esattamente questo: solo che lo fa senza che si possa dire da prima quale voto pesa di meno e quale pesa di più. Quindi, una tensione c'è. Si avverte la necessità di bilanciare il valore del voto uguale con il principio della governabilità, che pure può intendersi come costituzionalmente protetto. Esiste una tensione tra rappresentatività e governabilità

Quindi, il fatto che si vada o meno ad un cambiamento forte del sistema politico è una scelta dello stesso sistema politico, della libera evoluzione delle forze che ne fanno parte. Non è una armatura giuridica che il legislatore

a quella di oggi, soprattutto a quella degli ultimi anni, anche relativa alla manipolatività eccessiva di alcuni quesiti referendari - rende oggi possibile che si abbia una pronuncia nel senso dell'inammissibilità del *referendum*. Non voglio dire cosa la Corte debba o non debba fare. Non spetta a me

Nell'intenzione dei proponenti dovrebbe ridurre la frammentazione del sistema politico, dovrebbe semplificarlo. Attenzione: lo dicevano già nei primi anni

facilissimo, infatti, fare un listone unico in cui confluire e il giorno dopo le elezioni tornare a separarsi. Io oggi faccio parte di una piccola forza politica - anche se penso e spero che sarà grande molto prima delle elezioni - e non sono affatto preoccupato del passaggio referendario. Il mio potere contrattuale non me lo

in equilibrio. Le forze politiche sono ovunque frammentate. Le assemblee elettive sono rissose. I Governi non sono efficaci. Non siamo governati meglio. Al contrario. Per questo noi proponiamo il modello tedesco, diciamo, come migliore

Io dico che dobbiamo avere più rappresentanza: la decisione politica è difficile, certo, ma bisogna capire perché. Ne abbiamo visto ieri,

di cose fatte bene e di molte cose fatte male su questo tema che, a dire la verità, hanno interessato la prima e la seconda Repubblica, perché non è vero che la prima Repubblica non abbia dato un contributo. La legge sulla quale noi abbiamo basato la vita di tre legislature, la prima, la seconda e la terza della seconda Repubblica, fu approvata nel corso della prima, il cosiddetto *Mattarellum*. I tentativi di cambiamento elettorale che sono intervenuti per meglio perfezionare quel provvedimento sono stati più di uno. Alcuni hanno persino persino mobilitato la metà del corpo elettorale del Paese: ricordo il *referendum* che non ottenne il 50 per cento perché ci eravamo dimenticati di aggiornare le liste elettorali e abbiamo contato anche quelli che erano nel frattempo passati ad altra vita tra gli elettori attivi, perché altrimenti quel *referendum* avrebbe avuto un consenso straordinario e un effetto di cambiamento della legge che avrebbe sicuramente segnato un passaggio importante per il sistema politico. Vi è stato un tentativo in Parlamento, nella legislatura 1996-2001, andato molto avanti nella discussione qui al Senato in prima Commissione - presieduta dal senatore Villone - che si fermò non perché non c'era un accordo di maggioranza sulla legge da fare. Si fermò perché l'opposizione accese il semaforo rosso e ci disse: non possiamo attuare la riforma elettorale, se non siamo tutti d'accordo; e poiché non siamo d'accordo, la riforma elettorale non si deve fare! In quella occasione la maggioranza di allora, di centro-sinistra, valutò, pur avendo i numeri, che non fosse opportuno cambiare la legge elettorale, in assenza di un largo consenso. Ed arriviamo così alla legge "porcata", come l'ha definita il suo principale protagonista. Sono stato testimone in Commissione, prima alla Camera, di tutti i passaggi e devo pur che il vero protagonista di quella legge, nella fase propositiva e nella soluzione di tutti i passaggi complicati che ha dovuto attraversare - bisogna dare onore al merito - è stato l'allora ministro Calderoli, l'attuale Vice presidente dell'Assemblea cioè, che si adoperò in ogni circostanza, quando nascevano problemi in quella maggioranza, che si rifiutò di avere un rapporto con l'opposizione di allora smussare gli angoli, e quindi a definire nella maniera più precisa la "porcata" finale, come l'ha definita lui, sulla quale poi si votato. votato. Se affrontiamo questa discussione senza avere chiaro da dove veniamo, questo è il primo errore grave politico che possiamo commettere. Dobbiamo avere tutti scienza e coscienza di quanto abbiamo fatto e detto, su cui ci siamo impegnati. secondo elemento politico che si deve tenere presente è che non stiamo discutendo di legge elettorale - diciamo la verità - perché siamo tutti convinti che sia così urgente! Due fatti segnano l'urgenza: il primo è che vi è stato un gruppo di cittadini, tra i quali ci sono anche io, ed autorevoli professori che hanno studiato la Costituzione (e che probabilmente potrebbero loro fare lezione a noi e non noi a loro su questa materia perché essa e' stata

L'altro fatto politico che determina l'urgenza è, ahimè, un fatto negativo: siamo appena ad un anno di vita di questa legislatura ed abbiamo già attraversato una crisi di Governo. E all'indomani di questa crisi di Governo, autorevolmente, il Presidente della Repubblica ha fatto presente a tutti noi che non si può andare ad elezioni, anticipate ma non solo, se non si cambia la legge elettorale. Questi sono i due fatti politici rilevanti. Ve ne sono poi anche altri vari ed eventuali che non richiamo, che costringono l'urgenza e ci impegnano a sviluppare una iniziativa in questa direzione. allora che questi elementi di contorno politico ci devono aiutare a sviluppare una discussione di merito, sapendo che non esiste una legge elettorale perfetta e che non ci possiamo avventurare troppo sui modelli tedesco, spagnolo e quant'altro perché siamo in Italia ed è bene che piantiamo le radici qua, anche sulla base dell'esperienza fatta finora; sapendo che i cittadini hanno bisogno di un segnale per superare la crisi nei confronti della politica, che non è una novità di questi giorni. Sono anni ormai che la politica è all'ultimo posto della classifica sul piano della fiducia: un sistema bipolare, seriamente e non apparentemente tale; un rapporto tra cittadini ed eletti, che deve essere assolutamente diverso da quello che abbiamo registrato,

Infine, la coesione e l'affinità programmatica, perché abbiamo purtroppo bisogno di superare una difficoltà nel nostro sistema politico, soprattutto se lo paragoniamo agli altri. Non possiamo infatti guardare alla Francia

in maniera così efficace. Non abbiamo presentato una proposta di legge come Gruppo dell'Ulivo. Pensiamo in questo modo di aver contribuito a creare un clima che trovi un consenso fondamentalmente sui princìpi che adesso ho indicato.

Quando discutiamo di legge elettorale esiste il Parlamento, esistono i Gruppi che lo rappresentano e ovviamente, siccome operiamo tutti nella politica, ciascuno di noi si muove cercando di non frantumare quel po' di coesione esistente, semmai di rafforzarla e quindi di affermare un principio bipolare, che, seppur pieno di cerotti e ferite, ancora esiste e che noi vorremmo, al contrario, rafforzare cambiando la legge elettorale. *(Applausi

di avviare e aiutare un confronto tra le forze politiche di maggioranza e opposizione per definire una nuova legge elettorale, anche per corrispondere, ovviamente, a una precisa indicazione che ci è venuta dal Presidente della Repubblica. abbiamo dedicato alcune giornate di discussione, anche qui al Senato, alla presenza del rappresentante del Governo, il ministro Chiti,

delineare un cammino comune da percorrere, ma soprattutto un risultato finale che fosse di soddisfazione per i partiti di maggioranza e di opposizione. Eravamo ottimisti all'inizio, però dobbiamo dire con chiarezza che dopo la costituzione del Partito democratico alcune componenti del vecchio DS, soprattutto alcuni partiti politici (ricordo l'intervento di

Certamente dobbiamo prendere atto di questa difficoltà. Non mancheremo comunque di mantenere la nostra attenzione sul tema e ringrazio anche il senatore Calderoli, che è stato molto attivo nel tentativo di mettere insieme un po' tutti i *desiderata*, tutte le richieste, per cercare di pervenire a un nuovo sistema elettorale. elettorale. Continueremo a dare il nostro contributo, parteciperemo al dialogo. Non abbiamo fatto nostre proposte politiche, ma guarderemo con attenzione a quanto accade e daremo la nostra adesione. Questo è l'impegno politico di Alleanza Nazionale, a due condizioni, Presidente, colleghi: in primo luogo, che si consolidi il bipolarismo; in secondo luogo, che si arrivi a un sistema elettorale per il quale sarà il cittadino a scegliere la classe politica, la classe dirigente che dovrà governare il Paese, prima e non dopo. A queste due condizioni esamineremo le proposte che verranno fatte, altrimenti c'è il *referendum* in atto, ai cui risultati guarderemo con grande attenzione.

quella cioè che è stata indicata dal senatore Calderoli, mi pare in accordo con la stessa Commissione. Metto ai voti

segnalare che stamani il TG1 in tutte le sue edizioni ha aperto il notiziario dando un'informazione gravemente scorretta, oserei dire falsa. Il telegiornale - mi scusi, signor Presidente, se richiamo la sua attenzione - ha aperto dicendo che ieri sera il Senato ha approvato l'ordine del giorno della maggioranza che «approva l'operato

sa bene, come sanno i colleghi, che questo non è vero, tant'è che ieri sera il presidente Marini ha espresso con chiarezza che il Senato aveva approvato l'ordine

aveva riferito con precisione e correttezza quanto era avvenuto in quest'Aula; evidentemente questo non era piaciuto a qualcuno e stanotte una manina ha sostituito la cronaca veritiera con quella falsa. falsa. Ritengo che il Senato avrebbe diritto di godere del rispetto delle sue deliberazioni (che piacciano o no). Posso comprendere che il servizio pubblico e il TG1 abbiano un orientamento filogovernativo,

Chiedo quindi l'intervento della Presidenza del Senato, perché il servizio pubblico ristabilisca la verità dei fatti. *(Applausi

sarò brevissimo, telegrafico. Sulla stessa lunghezza d'onda del collega...

Commissione. Vorrei quindi invitare i segretari d'Aula, i collaboratori della Presidenza a tener conto di questo. Vorrei aggiungere che, se mi fosse stata data la parola prima del voto sull'ordine del giorno della maggioranza, non si sarebbe verificata quella *bagarre* sull'ammissibilità della seconda parte di quell'ordine del giorno, perché era evidente che tale ordine del giorno era inammissibile perché contrastava con degli ordini del giorno già bocciati dall'attuale maggioranza. **Sulla

il Senato non si riunirà e nel frattempo sarà presente in Italia il presidente degli Stati Uniti d'America, George W. Bush.

la prima volta, a sua Santità Benedetto XVI, ma che ha sentito il dovere di intrattenersi anche con le autorità italiane. Il nostro ringraziamento per gli Stati Uniti d'America trova proprio in questo anno e in questo mese il sessantesimo anniversario del piano Marshall, al quale l'Italia deve molto per la sua ricostruzione democratica, civile, economica e sociale. Con gli Stati Uniti d'America siamo impegnati, in questo momento, in varie missioni militari, in particolare in Afghanistan, per la lotta contro il terrorismo, quindi riteniamo di avere dei doveri e dei diritti nei confronti degli Stati Uniti d'America.

elementi tali da suscitare un'approvazione al saluto e al ringraziamento che dobbiamo dare agli Stati Uniti d'America per il loro impegno nel mondo. Devo anche osservare, signor Presidente, che trovo alquanto strano che capi dei partiti che fanno parte della maggioranza vadano in piazza probabilmente per protestare contro il Presidente degli Stati Uniti. Naturalmente, credo che il diritto di riconosciuto a tutti i cittadini, ma che lo facciano responsabili dei partiti che sostengono la maggioranza di un Governo che collabora in punti essenziali del nostro programma con gli Stati Uniti d'America lo trovo alquanto strano. In ogni modo, desidero esprimere il nostro impegno per la collaborazione con gli Stati Uniti d'America e con il suo Presidente, con il saluto più cordiale che rivolgo a nome del mio Gruppo e, credo, a nome di tutti i Gruppi della Casa delle Libertà, che è diretto con il cuore, col sentimento e anche con rispetto politico.

che, modificando la lettera *c*) dell'articolo 1, prevede che si sospenda per un mese l'attività dell'unità produttiva nell'eventualità in cui si accerti che in quella stessa unità produttiva sia occupato almeno un lavoratore irregolarmente soggiornante. Il problema che mi ero posto, e che avevo rappresentato al Presidente chiedendogli cortesemente di intervenire, era questo: quando siamo in presenza di una unità produttiva, com'è nella stragrande maggioranza dei casi in questo Paese, con quattro, cinque, sei dipendenti

diamo la stura alla possibilità di chiudere numerosissime e piccolissime aziende solo perché, probabilmente, verrà accertato che, in una di quelle piccole aziende con

norma poco fa approvata non può non avere conseguenze sul piano generale in riferimento all'articolo 1, dove già era previsto un aggravamento della pena nell'eventualità vi fosse un solo

che il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto e con una sanzione di 5.000 euro per ogni lavoratore quando abbia alle sue dipendenze più

ma nel farlo mi pare non tenga davvero conto delle ragioni dei lavoratori. Non mi riferisco al lavoratore irregolarmente soggiornante, ma a quei cinque lavoratori assolutamente in regola ai quali deriverà un inevitabile danno da questo vostro furore legalistico, che aveva un senso quando i lavoratori erano tre, ma che non può averlo quando il lavoratore è uno e quindi assolutamente marginale rispetto alla struttura sia pure minimale di un'azienda. Spiegatemi poi la ragione per la quale, quando si si tratta di un datore di lavoro diverso, si sanziona il datore di lavoro che - parliamoci chiaro - sfrutta il lavoratore irregolarmente soggiornante tanto quanto l'organizzazione che lo recluta, perché è lui che lo assume. Ebbene, per quel datore di lavoro voi prevedete esclusivamente la pena dell'arresto, quasi che vi possa essere un'organizzazione tesa al reclutamento e allo sfruttamento dei lavoratori stranieri senza che vi siano datori di lavoro che assumono

che i lavoratori irregolarmente soggiornanti possano assumere una attività lavorativa in Italia e conseguentemente irrogate una serie di sanzioni a destra e a sinistra, senza guardare in faccia nessuno. Potete farlo,

nel Testo unico sull'immigrazione, e in particolare dall'articolo 22, comma 12, tanto che la prima disposizione sulla quale interviene in senso modificativo l'articolo 2 è proprio il comma 12 dell'articolo 22. Qual è la particolarità dell'intervento di rettifica? La prima parte del comma 12 è uguale a quella contenuta nel Testo unico sull'immigrazione. C'è però un'aggiunta. In sostanza, mentre l'irregolare occupazione di stranieri clandestini, in termini generali, trova la sanzione dell'arresto da tre mesi ad un anno, cui si aggiunge l'ammenda di 5.000 euro, vi è una sanzione inferiore se il datore di lavoro è persona che ha bisogno di collaborazione familiare o domestica. In questo caso, si prevede la sola ammenda di 4.000 euro. Trovo incongruo che in un provvedimento che vuole essere più incisivo contro lo sfruttamento di lavoratori irregolari vi sia una sanzione graduata che il datore di lavoro sia un imprenditore o un padre di famiglia, o comunque una persona che ha bisogno di collaborazione nella propria casa. In realtà, incongruo non è se questa aggiunta viene inserita nel quadro di ciò che l'attuale Governo, con il sostegno intermittente dell'attuale maggioranza, ha fatto nell'ultimo anno e, in particolare, con quel provvedimento abnorme che ha riaperto i termini del decreto sui flussi del 2006 e ha trasformato un decreto sui flussi, integrativo (quello che ha seguito l'originale testo del 2006), in una sostanziale sanatoria.

tant'è vero che si è fatto un giro abbastanza contorto per evitare che costoro tornassero a casa e fingessero di venire in Italia per la prima volta regolarmente, facendosi rilasciare un visto e seguendo la procedura prevista dal Testo unico sull'immigrazione. In questo contesto,

poiché gran parte di quella sanatoria di fatto è stata adoperata per il lavoro domestico, il datore di lavoro non può essere punito addirittura con la pena dell'arresto, cui si aggiunge l'ammenda, ma con la sola ammenda. Logica e coerenza avrebbero voluto che, se avete fatto una sanatoria per i per i lavoratori stranieri, la faceste anche per i datori di lavoro che si trovano in questa condizione; invece, vi accontentate sempre delle soluzioni intermedie, un po' come è accaduto ieri in quest'Aula: cacciate via il generale Speciale, ma, in via intermedia, sospendete le deleghe al vice ministro Visco. Mi sembra che quella adottata con il nuovo comma 12 sia una soluzione intermedia che non so quanto soddisferà. Certo, nella prospettiva di una maggiore chiarezza, avrebbe giovato che (come noi abbiamo fatto con la regolarizzazione di cinque anni fa, una regolarizzazione reale, cioè seria, che che passasse formalmente da atti coerenti) vi fosse stata una esenzione dalla sanzione anche per il datore di lavoro. L'articolo 2 presenta un secondo aspetto veramente singolare che non posso fare a meno di sottolineare, cioè il nuovo comma 12-*ter* che viene inserito nel Testo unico sull'immigrazione. Cosa prevede questo nuovo comma? Prevede che «il luogo di lavoro», leggo testualmente, «ove sia occupato da un lavoratore straniero che versi nelle condizioni di cui al comma 12-*bis* può essere sottoposto al sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale». Vorrei capire da chi ha scritto questa norma (e deve averci pensato, mi auguro, prima di scriverla) quale ne sia il senso. Se esistono, in qualsiasi caso specifico, le condizioni per applicare il sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, non vi è necessità, ogni qual volta ricade una fattispecie concreta per applicare questa disposizione cautelare reale, di scrivere che va applicata: essa vale in termini generali. Pertanto, se vi è un'azienda, o comunque un luogo, dove sono occupati lavoratori stranieri clandestini, e quindi vi è occupazione irregolare che necessita, sulla base dei criteri che rendono applicabile il sequestro preventivo, l'irrogazione concreta di tale misura cautelare, non vedo perché si senta la necessità

di manzoniana memoria, gride che si ripropongono non soltanto, sul piano sostanziale con questo inutile, confuso, contraddittorio e per certi versi dannoso, nell'applicazione concreta che può avere, articolo 630-*bis* del codice penale, ma anche nelle misure cautelari reali che si vogliono introdurre a sostegno di questa norma. Credo sia un ulteriore sintomo che dovrebbe far riflettere l'intero Senato sulla inutilità - e già così andrebbe bene - e la dannosità di questo provvedimento.

termine si riferisce ad una condizione particolare. Non parliamo di un lavoratore irregolarmente presente, che lavora e magari è pagato in nero;

devono ricorrere (non nella condizione di lavoro, perché se la condizione di lavoro fosse quella del lavoro forzato avrebbero la stessa pena) a certe modalità di accesso alla manodopera. Abbiamo pertanto ritenuto giusto - e la rivendico come una scelta giusta - non sottoporre le famiglie a quella stessa condizione, proprio per i difetti che derivano, anche dal punto di vista della politica, dell'estendersi dello Stato sociale. Tale è la questione di cui parliamo. I flussi migratori e le modalità inerenti sono altra questione. Noi parliamo di come si sanziona il lavoro forzato, che - ricordo

di un punto preciso in cui il mercato criminale incontra il mercato legale, che spesso è quello dell'impresa e della riduzione al lavoro forzato.

- ripeto l'intervento perché il Governo, a mio parere, è ancora in tempo - il provvedimento si connette in maniera maldestra alla volontà del Governo, che dovrebbe avere il diritto di governare se ne ha i numeri, la capacità, se non incede nell'arroganza e nella violenza come fatto nei giorni passati e soprattutto ieri e ieri sera; ciò qualora il Governo facesse dei provvedimenti, nel suo diritto di governare, coerenti tra loro. In Commissione bilancio abbiamo argomentato che il provvedimento si connette male è incoerente rispetto alla Amato-Ferrero. Sia la sottosegretario Lucidi che il vice ministro Danieli, nella precedente seduta, erano stati molto attenti alla

e che, come annunziato, sarà presentato alla Camera, e visto che questo provvedimento è soltanto in prima lettura in questo altro ramo del Parlamento, alla Camera si avrà probabilmente la lettura contemporanea della

caporalato. Torno sul tema perché la fretta di approvare un provvedimento che incentri l'attenzione del Governo sulla modifica degli articoli del codice penale attinenti e relativi allo sfruttamento dei lavoratori italiani e stranieri ha fatto nascere un articolato (anche se semplice, perché costa di due soli articoli) che non rispetta assolutamente la legalità, né la necessità di proporzionalità cui il legislatore

non regolarmente presenti sul territorio, si ha una pena inferiore rispetto a quella che vi potrebbe essere nei confronti di un datore di lavoro organizzato sotto forma di impresa che abbia la presenza di un solo lavoratore.

la necessità che l'organicità della produzione legislativa non possa essere violentata da una puntuale e disorganica riscrittura del codice penale.

infatti delle connotazioni di disparità di trattamento e quindi di incostituzionalità. La molteplicità delle osservazioni fatte da altri colleghi - e che continuo a fare

della maggioranza, a quella più estremistica e che vuole coprire la propria inefficienza con una pretesa di riguardo e di garanzia dei lavoratori stranieri,

dei lavoratori, ma anche del diritto di impresa, che non sia vessatoria e persecutoria nei confronti di chi in questo Stato lavora non soltanto per sé stesso, ma per garantire quel progresso che ci sembra

Presidente, ho sentito parlare poco fa di lavori forzati, quasi di riduzione in schiavitù. quindi riportare il discorso sulla reale dimensione del fenomeno e sui meccanismi che questa legge attiva.

e la violazione di altre norme. Invito il relatore a riflettere su quanto sto dicendo. Sostanzialmente, con queste norme applicate una legge quanto mai dura a favore dei lavoratori irregolarmente soggiornanti. Vorrei chiedere al relatore: nel caso in cui ci si trovi di fronte a lavoratori non irregolarmente soggiornanti, ad esempio a lavoratori italiani che lavorano in una microimpresa italiana,

di una sorta di pregiudizio legislativo negativo discriminante nei confronti dei lavoratori italiani: se in queste stesse condizioni si trova un lavoratore italiano, la normativa non prevede né la chiusura dell'impresa, né il sequestro del luogo di lavoro.

sia un lavoratore extracomunitario immigrato irregolare e non nel caso in cui ci sia un lavoratore di nazionalità italiana? Perché nell'ultimo Voi sapete benissimo che non solo nel Sud, ma anche e soprattutto nel Centro-Nord, questo tipo di rapporto irregolare di lavoro è una costante. Non riesco a capire perché, allora, nei confronti di un lavoratore italiano non si debba parlare di lavoro forzato,

inquadrati e lavoratori che presentino questi *standard* di tassatività per la fattispecie delittuosa del grave sfruttamento, allora potremo ragionare, ma perché discriminate con questa legge tra lavoratori di nazionalità italiana e lavoratori irregolarmente soggiornanti?

che non si rendono conto nemmeno di cosa legiferano e di cosa decidono: a futura memoria, tra l'indifferenza - ne prendo atto dei colleghi della sinistra, perché evidentemente il lavoro forzato è applicabile agli italiani e non agli irregolarmente soggiornanti, ho voluto sottolineare questo fatto perché in futuro un cronista potrà anche chiedersi perché queste leggi in difesa dei lavoratori irregolarmente soggiornanti non erano applicabili nel caso

che indicano presunte contraddizioni all'interno del testo e anche interferenze rispetto al discorso più generale e agli orientamenti che emergono dal disegno di legge

anche da indagini apposite. Il fenomeno è particolarmente serio proprio nei confronti di soggetti immigrati: quei clandestini che arrivano nelle condizioni drammatiche, che purtroppo ci vengono rappresentate quotidianamente, sono quasi tutti vittima di di organizzazioni che fanno intermediazione illegale e molto spesso violenta. Quindi, è su questo che concentriamo l'attenzione prevedendo, non solo

che ha una sua autonomia. Per questo abbiamo voluto insistere rispetto al discorso generale di contrasto all'irregolarità nell'immigrazione. Riteniamo che la gravità del fenomeno richieda

si presti molto all'irregolarità. Sull'aspetto generale, comunque, c'è un piccolissimo intervento che andrà certamente ripreso e completato quando si affronterà il tema generale o il disegno di legge governativo sull'immigrazione.

che caratterizza l'intero provvedimento: l'essere avulso rispetto ad una più generale revisione della disciplina relativa ai flussi migratori e soprattutto a quelli di essi che hanno carattere di irregolarità.

Questa separazione fra i due provvedimenti si evidenzia poi nella pesante asimmetria che si può riscontrare

si confondono con fattispecie già presenti e già significativamente sanzionate dall'attuale ordinamento e il fortissimo ridimensionamento delle sanzioni relative invece ai clandestini stessi. Tanto che noi pensiamo che il disegno di legge governativo di modifica della recente legge Bossi-Fini avrà l'effetto di attrarre flussi di clandestini, nel momento in cui ipotizza una serie di disposizioni che sembrano tutte orientate a voler difendere il cittadino clandestino dalle istituzioni pubbliche italiane, anziché difendere il nostro ordinamento da quei da quei flussi clandestini che sono destinati a sovvertire significativamente la nostra stessa coesione sociale. Credo che queste disposizioni siano poi spesso caratterizzate da una significativa sproporzione tra il reato ipotizzato e la sanzione stessa. Ha opportunamente ricordato poco fa il collega Nitto Palma quanto sia assurda la sanzione che consiste nella cessazione forzosa dell'attività, una sanzione che ritorna in più provvedimenti proposti dal Governo. Lo stesso disegno di legge che verrà all'esame di quest'Aula

sospensione dell'attività dell'unità produttiva, con danno verso terzi incolpevoli, come certamente sono gli altri lavoratori dell'impresa. non tiene conto nelle attività produttive di quel ciclo biologico del quale giustamente ci si preoccupa per le attività agricole, ma che non di meno caratterizza anche le attività più più generalmente produttive di beni o di servizi che hanno loro cicli che una volta interrotti possono produrre un danno irreparabile

conseguente alla forzosa sospensione dell'attività stessa. Il provvedimento quindi seguire un approccio quasi ideologico. Anche quando si preoccupa di contrastare il caporalato, non posso non rilevare l'ulteriore asimmetria tra l'inasprimento delle sanzioni nel caso di esercizio abusivo abusivo dell'attività di intermediazione di manodopera e il diffuso atteggiamento di tolleranza da parte delle delle istituzioni nei confronti di varie forme di esercizio abusivo dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Penso a quei molti siti che ancora impunemente offrono questo servizio, penso perfino ad attività paraistituzionali: non so se più recentemente abbia regolarizzato la sua posizione un consorzio universitario che si occupa di promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La legge Biagi aveva ampliato la possibilità di esercitare questa funzione rispetto al monopolio di fatto che in passato si era mantenuto in capo ai centri pubblici per l'impiego, ma nel contesto di rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi per poter svolgere questa delicatissima delicatissima attività di intermediazione. Ma noto che vi è uno strano atteggiamento di tolleranza verso le moltissime attività abusive che, come ho detto, sono consentite anche dalla rete e che la rete favorisce ancor più o che talora sembrano sembrano trapelare anche da determinati annunci sugli organi di informazione, salvo poi, nel caso del lavoratore clandestino, ricorrere appunto ad ad un inasprimento dalle sanzioni penali, come se questo tipo di irregolare funzione non dovesse rilevare, anche quando si esercita nei confronti di lavoratori non clandestini, regolarmente presenti nel nostro Paese o perché residenti o perché regolarizzati. Insomma, come al solito si agisce secondo una logica occasionale, cercando di incontrare magari una specifica emozione, che si definisce anche opportunamente in rapporto a determinate patologie, ma senza un approccio organico tendente a creare una situazione davvero di ordine effettivo per quanto riguarda i flussi migratori e quel contrasto più complessivo della clandestinità che chiediamo di realizzare anche a prevenzione dei

perché altrimenti non possono definirsi quelle attività di revisione delle quote d'ingresso nel Paese che si definiscono in relazione alle domande presentate, cioè a sanatoria delle domande di tutta la pressione migratoria che si è determinata attraverso la presenza effettiva già nel nostro Paese. Occorre spezzare questo circolo vizioso applicando fino in fondo la legge Bossi-Fini e non pensare di rivederla nei termini già proposti dal Governo,

il lavoro delle Commissioni riunite non è stato inutile e tutto sommato si è raggiunto un buon risultato rispetto al testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo pervenuto al Senato.

sono originariamente forieri di confusione - voglio adesso definirla così ma la illustrerò meglio in questo mio breve intervento

un disegno di legge delega per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; quindi, stiamo discutendo in un contesto più ampio che è sorto da un sentimento comune e generalizzato per l'esplodere di una certa recrudescenza degli infortuni sul lavoro in

Per questo motivo, esiste una confusione anche nei tentativi emendativi di questo disegno di legge e il lavoro delle Commissione riunite comunque

all'interno della legge Bossi-Fini sull'immigrazione con una modifica sui cui princìpi ovviamente non posso che esprimere

assumendo posizioni molto particolari rispetto alla tutela del lavoro ordinario o alla

così nel testo originario) chi clandestinamente risiede nel nostro Paese e viene, in maniera orribile, sfruttato da qualche imprenditore di poco senso, poco senso, tutelando o incentivando la reazione a questo tipo di sfruttamento (come era previsto con il permesso di soggiorno, che invece nel testo proposto dalle Commissioni riunite non lo è più), non si risolve il problema.

Oltretutto, si creano anche delle disparità, per cui un lavoratore italiano che venga sfruttato, lavorando nel sommerso (quindi senza

viene sfruttato un extracomunitario clandestino, sa che le pene riguardanti il proprio datore di lavoro saranno inferiori a quelle

per avviare la diversa disciplina sanzionatoria dell'articolo 2, ma si sono trasformate, dal testo d'iniziativa del Governo a quello delle Commissioni

è un atto di violazione delle nostre leggi. Non si può pensare che sia esclusivamente una condizione subita, come può accadere ad esempio

A me dispiace che il senatore Ferrara esprima una opinione diversa dalla mia, tutto è legittimo, ma credo di avere almeno in questo momento la responsabilità della Presidenza dell'Aula che cerco di governare e di guidare nel modo più imparziale possibile. Se il senatore Ferrara intende intervenire sull'emendamento può farlo benissimo, ovviamente soltanto in dissenso perché per il suo Gruppo è iscritto a parlare in dichiarazione di voto il senatore Palma.

che i senatori dall'altro lato dell'Aula abbiano plaudito al suo intervento nei miei confronti, quello sì, mi dispiace perché hanno interpretato male il mio intervento, e mi dispiace

Non riesco a capire se la mia povera nonnina potrebbe inavvertitamente compiere un reato che possa rientrare in queste sanzioni penali o disciplinari. Infatti, potrebbe anche capitare che non conoscendo perfettamente le leggi che emana il Parlamento italiano, dato il grande bisogno di assistenza, trovandosi una persona dall'aspetto civile e bonario, disposta a dare una mano nelle faccende domestiche, anche attratta da un aspetto umano di reciproca assistenza e scambio di bisogno, possa non dico assumere, perché è un termine pesante,

corrispettivo di piccoli lavori domestici. Mi sfugge se in questo caso mia nonna rientra nella prima parte dell'articolo 2, che prevede

gli evasori in primo luogo, che probabilmente mettereste al rogo se questa pena fosse ancora prevista dal codice penale, come chi sfrutta i poveri soggetti provenienti da aree - ahimè - meno fortunate delle nostre, e forse dovremmo anche sentirci in colpa perché gli squilibri del mondo devono sempre, in ogni caso, avere delle responsabilità.

che probabilmente deve la sua magnificenza e le sue bellezze storiche, artistiche e architettoniche ad un unico fatto: per secoli e secoli ha soltanto sfruttato categorie sociali che avevano sicuramente molto meno diritti di quelle dominanti, anzi si può parlare proprio di autentica schiavitù. Vorrei sentire qualcuno che oggi inneggia a questa legge criticare e vergognarsi per quanto è stato fatto in questo Paese: mi sembra tutt'altro. Vanno ad esasperare gli aspetti del nostro patrimonio storico e artistico e, se vogliamo proprio

allora a riformulare un quesito di carattere generale che finora non ha avuto alcun seguito, perlomeno nessuno soddisfacente. L'intero disegno di legge, e quindi anche la parte di cui stiamo discutendo, proviene come fonte dal Governo e si sovrappone, lo ripeto per l'ennesima volta, ad una parte del disegno di legge cosiddetto Ferrero-Amato che il Consiglio dei ministri ha licenziato il 24 aprile di quest'anno. Abbiamo saputo dalle fonti di informazione che tra qualche giorno, in particolare il 15 giugno, sarà portato all'esame della Conferenza unificata Stato-Regioni, quindi esiste, esiste, non soltanto come testo varato dal Consiglio dei ministri ma come testo che sta conoscendo il suo *iter*: non è arrivato formalmente in Parlamento perché sono necessari questi passaggi, ma quando saranno completati arriverà. Il comma 1 del disegno di legge Ferrero-Amato delega il Governo ad adottare, entro un certo termine, una riforma integrale del Testo unico sull'immigrazione, senza nessuna eccezione di settori o di voci, ispirata ad una serie di principi e di criteri direttivi. Tra questi, la lettera *q)* del comma 1 dice: «favorire una adeguata tutela delle vittime di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, delle vittime di tratta,» e la virgola, in un testo di legge, ha carattere disgiuntivo e quindi alternativo rispetto a tutte le ipotesi in discussione, «delle vittime di violenza o grave sfruttamento». Mi fermo qui perché questo termine, questo aggettivo e questo sostantivo, «grave sfruttamento», costituiscono il fulcro attorno a cui ruota il disegno di legge che stiamo discutendo, perché l'articolo 603-*bis* che si vuole introdurre e che abbiamo già esaminato in sede di discussione dell'articolo 1 di questo disegno di legge ha come condotta centrale, come elemento qualificante ed essenziale, il grave sfruttamento dei lavoratori, di qualsiasi tipo di lavoratore, non soltanto quelli extracomunitari. Su questa voce

Il Governo dovrebbe darci una spiegazione logica, giuridicamente convincente, derivante dalla comparazione tra l'uno e l'altro disegno di legge di provenienza del medesimo Esecutivo che escluda che vi sia ciò che invece è evidente, cioè una ripetizione di norme. A completare un quadro che uno psichiatra definirebbe schizoide, provvede poi il Ministro della solidarietà, il quale in un'ANSA del 4 giugno, annuncia testualmente: «Chiederò a Romano Prodi un decreto-legge che attui già per questa estate la revisione dell'articolo 18», sottinteso della legge sull'immigrazione, «cioè la possibilità per il lavoratore straniero al nero di denunciare il datore di lavoro ottenendo in cambio il permesso di soggiorno». Aggiunge il ministro Ferrero, sempre sulla base di ciò che dice l'agenzia ANSA: «Siccome il disegno di legge di revisione dell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione è fermo al Senato, occorre evitare che anche questa estate si riproduca questa situazione vergognosa per cui i datori di lavoro agricolo continuano ad assumere in nero tanti lavoratori stranieri». Evidentemente le comunicazioni all'interno del Governo non funzionano al meglio, perché il ministro Ferrero non sa che da circa due mesi non stiamo discutendo più della modifica dell'articolo 18 del Testo unico dell'immigrazione, bensì di un'altra cosa che parte da quel riferimento normativo ma che ha raggiunto, per lo meno nominalmente e formalmente, altre configurazioni. Ma questa è una ulteriore ragione per tentare di capire un esponente qualificato, cioè un Ministro che ha una delega specifica, purtroppo per l'oggetto della delega, nella materia dell'immigrazione, che fa parte di quello stesso Governo che dice che questo testo va bene e che deve andare avanti, sostiene invece che il testo è fermo, che il Senato non lo sta esaminando e che va superato con un decreto-legge, che sollecita al Presidente del Consiglio. Io vorrei capire qual è la posizione finale del Governo. il Governo può anche dire che si impegna a disporre lo stralcio. Poiché tutto quello che dice il Governo, a mio avviso, merita il massimo dell'ossequio - perché tutti gli impegni che assume poi vengono puntualmente onorati - ci accontenteremmo. Il Governo potrebbe dire in Aula che si impegna a disporre lo stralcio, in sede di discussione del disegno di legge delega di riforma dell'immigrazione**,** della lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1. Ma non lo fa. Anzi, conferma l'esistenza di due disegni di legge, approvati dallo stesso Consiglio dei ministri, che per una parte coincidono. Non si sa quale dei due prevarrà. E nel frattempo, un Ministro, con competenze specifiche nel settore, annuncia o chiede al Primo ministro un decreto-legge, che riporti nella versione originaria, presentata alle Camere, quella fondata sulla riforma dell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, il testo che oggi discutiamo. Mi permetto di dire al Governo: fermatevi e fateci capire che cosa volete fare! Sulla base delle indicazioni che darete al Parlamento, questo sarà nella condizione di poter operare, facendo un minimo di chiarezza. Fino a quando queste risposte non arriveranno, sarà difficile che questa chiarezza ci sia.

Le argomentazioni e obiezioni oggetto dei loro interventi onestamente non mi convincono e chiederei loro cortesemente di prestare, se vogliono, un minimo di attenzione al mio intervento per taluni problemi

così come non vi è dubbio che le sanzioni devono essere gravi e devono avere per ciò solo una loro forza deterrente. Qual è il problema che avevo posto prima? È un problema molto semplice: quando nell'iniziale norma si parlava di tre lavoratori e della sospensione dell'attività dell'unità produttiva, sostanzialmente il legislatore fissava un tetto presunto di illegalità, dal quale fare scattare una determinata sanzione. Questo tetto di illegalità è retrocesso all'occupazione di un solo lavoratore dipendente.

una anomala situazione di responsabilità oggettiva, ormai straniera nel nostro ordinamento, anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale che vi è stata con riferimento ai rari casi di responsabilità oggettiva ancora esistenti nel nostro sistema penale. Perché dico questo? Per un motivo molto semplice: la legge dovrebbe essere un sistema completo. Dovrebbe, comunque, tentare di esserlo. Il vostro è un sistema incompleto, direi gravemente incompleto. La domanda che pongo al relatore, al senatore Zuccherini e, se mi è consentito anche all'onorevole rappresentante del Governo, onorevole Lucidi, è la seguente: il datore di lavoro che assume un dipendente proveniente dall'organizzazione criminale di cui all'articolo 603-*bis* di quale pena risponde non concorrendo nel reato? nel reato? Voi non avete previsto un'autonoma fattispecie di reato per il datore di lavoro che assume quel tipo di dipendente.

Onorevole Lucidi, colleghi senatori, il dato è inequivocabile proprio scorrendo l'articolo 2, ove avete inserito

lettera *b)*, istituiva dell'articolo 12-*bis*, con la quale sostanzialmente dite che il datore di lavoro che assume

reato questo sicuramente meno grave rispetto a quello di intermediazione di cui all'articolo 603-*bis*, sostanzialmente risponde di una determinata pena, e nel caso in cui evidentemente vi dovessero essere lavoratori di un certo tipo vi sarebbe un sequestro preventivo. Mi chiedo e vi chiedo, e vorrei una risposta sul punto: il datore di lavoro che assume dipendenti e lavoratori che provengono dall'attività di sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis* di quale pena risponde, se non concorre nel reato di cui all'articolo 603-*bis*? Poiché nel sistema penale, grazie a Dio, vige il principio di legalità e quello di tassatività per cui *nulla* *poena* *sine lege*, evidentemente ci troviamo di fronte a un comportamento che non è sanzionato penalmente e che, pur non essendo sanzionato penalmente, vede, come accessorio di una responsabilità senza colpa su un fatto non ritenuto illecitamente apprezzabile, la sospensione dell'azienda. Si potrebbe ragionare in modo diverso

Noi non abbiamo previsto - ma, ove mai l'aveste prevista vi chiedo di dirmi qual è la norma che sanziona questo particolare comportamento - la fattispecie del l'organizzazione, che a sua volta sfrutta e assume i lavoratori, quindi un soggetto che non concorre con l'organizzazione ma ne utilizza semplicemente i sistemi (se poi mi dite qual è la norma evidentemente il mio ragionamento salta). Se dovessimo

è comunque una forma sia pure più grave di intermediazione abusiva, per cui potremmo dire che il datore di lavoro verrebbe ad essere punito ai sensi della disposizione dell'introducendo articolo 12-*bis*.

quanto non previsto - del datore di lavoro con riferimento all'articolo 603-*bis*, prevedete il sequestro preventivo dell'azienda. Il che evidentemente equivale a dire nomina di un commissario e prosecuzione dell'attività dell'azienda.

è punito con la pena che volete), e allora possiamo anche rientrare nella legittimità della sanzione di cui alla lettera *c)*, oppure il sistema è destinato a saltare sotto il profilo costituzionale per una serie di ragioni.

perché il fatto è quello dell'organizzazione; inoltre, non prevedete nessuna possibilità di sanzione amministrativa, per comportamento illegittimo e illecito a carico del datore di lavoro che assume quel tipo di dipendente.

doveste immaginare che comunque sarebbe applicabile l'articolo 12*-bis* come forma generale all'interno della quale dovrebbe rientrare anche

alla Camera apporteranno le loro modifiche, oppure, se vorranno, non le faranno, ma sarebbe grave perché questa normativa è destinata a cadere davanti al vaglio della Corte costituzionale. Mi chiedo: non sarebbe forse opportuno

con riferimento all'articolo 2, introduca una fattispecie penale che riguarda quel tipo di lavoro. Siccome vedo qualche sorrisino, non è un intervento ostruzionistico. Vi invito a dirmi qual è la norma che punisce il comportamento del datore di lavoro che assume i dipendenti usufruendo dell'attività dell'intermediazione di cui alla fattispecie dell'articolo

mi asterrò dalla votazione di questo emendamento non perché non ne condivida il principio (già nella scorsa legislatura su iniziativa mia e di altri colleghi si era individuato nello sfruttamento del lavoro nero

È scritto male perché, quando si usa l'avverbio «contestualmente» con riferimento a «non più di due lavoratori» c'è un avverbio in più, cioè «contestualmente», perché la contestualità non può che riferirsi a due lavoratori, oppure ci sono tre parole in più, cioè «non più di».

perché questo potrebbe portare a dubbi interpretativi estremamente pericolosi, sia sotto il profilo della contestualità sia con riferimento al numero. contraddittoria se guardiamo la vicenda con riferimento alla posizione del lavoratore, perché la sanzione viene irrogata al datore di lavoro anche sotto forma di deterrente, come punizione con riguardo alla posizione di un lavoratore sfruttato in nero. Mi chiedo qual è la differenza tra un lavoro svolto tra le mura domestiche e uno svolto con lo stesso numero di ore presso un'impresa

vi è certamente una norma sanzionatoria inferiore che ritiene che quel tipo di lavoro in nero sfruttato sia meno importante rispetto ad ad altro tipo di lavoro. Non mi si venga a dire che comunque, mentre per gli altri tipi di lavoro sono previsti anche l'arresto e un'ammenda di 5.000 euro per il datore di lavoro, qui si pensa ad un lavoro tra le mura domestiche, perché evidentemente la differenza non esiste. Vorrei dire, infine,

nella confezione della sanzione che non ha ragione di essere, perché è una fattispecie semplice: due lavoratori contestualmente impegnati. Aggiungo l'entità della sanzione è veramente eccessiva per una famiglia: in questo modo non si colpiscono i ricchi: si colpisce anche la nonna del senatore Divina che ha una badante che viene la notte

da una famiglia e qui non ci stiamo riferendo a ceti medi o a ceti ricchi.

Vorrei rilevare che ieri in quest'Aula si è fatto un forte richiamo alle abitudini americane, si è parlato di Truman e di MacArthur, ma l'atteggiamento degli americani nei confronti degli immigrati non è certo quello che noi vogliamo introdurre con l'articolato in esame. Siamo, in verità, per una soluzione che sia adatta alla situazione italiana, perché l'Italia certamente soffre di una incapacità ad accogliere gli immigrati con i livelli istituzionali quali e contemporaneamente ha un problema del caporalato in campagna che probabilmente non è quello che esiste in America o in Inghilterra, visto che veniva richiamata anche la tradizione inglese. A parte il distinguo (i richiami andrebbero fatti con parsimonia, non in eccesso, perché l'Italia è l'Italia, l'America è l'America e l'Inghilterra è tutt'altra cosa rispetto alla stessa America e, in maniera più specifica e precipua, alla situazione italiana), noi non siamo contrari al provvedimento perché siamo a favore del caporalato: siamo contrari al provvedimento - è questo il distinguo rispetto alla dichiarazione del senatore Palma e quindi mi asterrò - perché siamo contro il caporalato, ma certamente non lo possiamo affrontare (non me ne voglia il relatore) con l'articolato così com'è, pieno di contraddizioni, in cui - ripeto - viene trattato il caporalato, o meglio la violenza nell'introduzione del caporalato, come fosse una rapina (perché quando si parla di una pena fino a otto anni è come se si trattasse di una rapina senza aggravanti). Ci rendiamo conto di quale elemento distorsivo nella

sta dando al contrasto di questo disegno di legge sciagurato in quest'Aula. Infatti, il mio Gruppo è tutto preso

un altro uomo della stessa Goldman Sachs: il signor Tommaso Padoa-Schioppa. Questo è dunque un Governo di banchieri. E un Governo di banchieri che cosa fa, in realtà?

che estorce a Capitalia e a Geronzi - Matteo Arpe, non a caso, poi è amico del signor Prodi - qualcosa come una buonuscita dai 50 ai 70 milioni di euro, cioè un centinaio di miliardi di vecchie lire. E sottolineo il fatto che qui, in questi giorni, in quest'Aula, da parte della sinistra non sia venuta nessuna indignazione verso questa autentica estorsione, mentre ci si indigna se un parlamentare come indennità percepisce lo stipendio di un magistrato di Cassazione, perché a questo siamo ridotti: non possiamo nemmeno aspirare allo stipendio di un magistrato di Cassazione.

diventa difficile. Intervengo in dissenso dal mio Gruppo, quindi dichiaro che mi asterrò sull'emendamento proprio perché, come ho ricordato anche negli altri interventi, questo provvedimento è partito da un'idea che poteva anche essere condivisibile diventando una cosa totalmente non condivisibile. La giusta La giusta punizione delle persone che in qualche modo sfruttano delle altre persone, in particolare nel campo dell'immigrazione clandestina,

Qui, invece, voi portate avanti due cose che divaricano in maniera assolutamente inaccettabile questa posizione di partenza. Da una parte, state portando avanti la futura legge cosiddetta Amato-Ferrero, che sostanzialmente apre le porte a tutti e fa entrare qualunque persona; dall'altra, fate questo provvedimento che accentua una parte della Bossi-Fini, che considerata nel contesto era assolutamente omogenea a tutto il ragionamento, la estrae e la fa diventare una cosa assolutamente inaccettabile.

possono succedere moltissime altre cose. Sapete benissimo che all'interno delle organizzazioni extracomunitarie clandestine ci sono fior di falsari che stampano documenti falsi a profusione, in quantità industriale. Pensate al povero imprenditore normale, in buona fede (oltre che alla nonna del collega Divina),

senza necessità di iscriversi preventivamente. C'è anche una *ratio* in tutto ciò, perché spesso il dissenso può nascere dalla dichiarazione di voto del collega. Quindi, la pregherei di assumere

non ho una visione muscolare della contrapposizione politica, La democrazia sulla base dei numeri prevede in che modo una parte politica possa affermare il suo pensiero sull'altra parte politica.

PALMA *(FI)*. Per essere chiari, ripeto, non ho una visione muscolare della contrapposizione politica, tanto meno qui in Parlamento dove, indipendentemente dalle diversità delle idee politiche, politiche, il reale obiettivo è comunque di approvare una legge che sia il più possibile priva di errori.

cioè sostanzialmente che non si prevedeva una sanzione penale per il datore di lavoro che aveva assunto lavoratori usufruendo dell'organizzazione criminale di cui all'articolo 603-*bis* il che poneva una serie di problemi costituzionali. Ho chiesto correttamente al Governo, al relatore e ai senatori della maggioranza di indicarmi se quello che affermavo era sbagliato

per approvare un articolo 2, e successivamente una legge, che contiene un errore talmente talmente grave da poter inficiare l'intero impianto della legge sotto il profilo della sintonia costituzionale. Allora, vorrei fare con molta tranquillità, con molta chiarezza, un discorso semplice:

andare avanti, voi porterete probabilmente a casa questo risultato, che sarà però zoppo perché inficiato da un grave errore (davvero errore (davvero non so quale vantaggio ne potrete avere perché subirete tutti gli svantaggi dell'applicazione di una legge sbagliata per le ragioni che abbiamo detto), sempre che ci arriviate, attesa l'ora, a questo tipo di approvazione;

nel senso di confutare la validità e l'opportunità del *mix* che si viene a creare tra articolo 1 e articolo 2 del disegno di legge in corso di approvazione.

argomenti di carattere penale come l'articolo 2, ma che comunque si inquadra nel *range* degli interventi mirati a rendere meno appetibile possibile l'orrenda abitudine da parte di qualcuno di sfruttare il lavoro clandestino.

che a questo punto si sommano alla disciplina sanzionatoria in senso stretto, arrecando non solo un danno - è giusto che sia così - nei confronti di chi si comporta in una certa maniera,

si prevede anche in questo caso una disparità di trattamento in senso restrittivo

una sospensione, un'interruzione nel momento in cui ci fossero dei reiterati tentativi o reiterate azioni che vanno nella direzione che questa stessa norma vuole impedire. Si può pensare che alla fine le sanzioni interdittive siano sempre escluse perché c'è un certo tipo di attività produttiva; il danno ovviamente e sarebbe molto grave - ma c'è comunque in un qualsiasi altro tipo di attività produttiva in cui, magari per un periodo di tempo di un mese, come è previsto dalla lettera *c*) dell'articolo 1, possa essere prevista la sospensione dell'attività interessata. Io penso che questi tre diversi punti su cui interviene il disegno di legge siano da un lato in contraddittorio l'uno con l'altro e dall'altro rivelino evidentemente un approccio alla deterrenza, con la la sospensione dell'attività produttiva, assolutamente difforme e, ripeto, riguardando solo i casi che concernono l'impiego di manodopera extracomunitaria irregolare, addirittura lesivi dell'interesse dei lavoratori italiani.

questa norma nel suo insieme è per un verso inutile e per altro verso dannosa. È inutile nella parte che ripropone il comma 12, perlomeno fino alle parole «per ogni lavoratore impiegato», perché - non riesco a comprendere la tecnica legislativa - è esattamente la stessa disposizione contenuta nel Testo unico sull'immigrazione che è in vigore. La seconda parte, invece, sulla quale ho tentato di soffermarmi in un precedente intervento, prevede una sanzione di minore entità quando il datore lavoro non è un imprenditore

è vero che si ipotizza una pena inferiore rispetto a quella di insieme, ma immaginiamo che l'anziana signora, stanca di aspettare le lunghe file che la pessima gestione del decreto flussi, realizzato da questo Governo, ha determinato, si rivolga ad una persona compiacente che offre la propria disponibilità per trovare una collaborazione alle proprie dipendenze. In quel caso, non ricadrebbe più nella sanzione prevista dalla seconda parte del nuovo comma 12 dell'articolo 22, ma nella sanzione prevista dal comma 12-*bis*. Questa anziana signora, cioè, verrebbe punita addirittura con le reclusione fino a tre anni e la multa fino a 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato; se è una persona che ha bisogno almeno di un doppio turno, la sanzione verrebbe ancor più aggravata. costituisca per un verso uno squilibrio rispetto al datore di lavoro imprenditore (per la parte di maggior favore) per altro verso sia una sanzione assolutamente spropositata rispetto all'entità del caso concreto, tanto più che tutto l'articolo 2 si muove esclusivamente nell'ottica di chi impiega alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari e non li sfrutta. In caso contrario, cadremmo nell'ottica sanzionatoria dell'articolo 1.

in un caso previsto dalla parte precettiva della norma penale in questione, i presupposti per intervenire con un sequestro preventivo (quello disciplinato dall'articolo 321 del codice di procedura penale), qualcosa osta in assenza di questa disposizione, cioè del comma 12-*ter*, all'applicazione concreta di una misura cautelare reale come il sequestro preventivo? È una domanda che continua a restare senza risposta e quindi continuo a non capire la necessità di introdurre questa disposizione specifica, cioè di dire che, quando vi sono le condizioni previste dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria può utilizzare lo strumento di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale. Qualcuno lo dubitava? Che necessità c'è di questa sottolineatura, che sembra andare nella direzione di forzare la mano al pubblico ministero e poi al giudice che dovrà decidere? Il comma 2 stabilisce che, nell'ipotesi di intermediazione abusiva di manodopera, si applicano le stesse pene accessorie previste per la più grave disposizione incriminatrice di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. In questo caso l'incongruenza è totale. Se infatti in una ipotesi conclamata ed accertata di grave sfruttamento può trovare una ragione concreta l'applicazione di sanzioni accessorie davvero pesanti, che giungono (nell'ipotesi, riformulata con l'emendamento accolto, di sfruttamento, per esempio, anche di un solo lavoratore straniero) straniero) alla sospensione dell'attività dell'intera azienda per un mese, colpendo quindi anche gli altri incolpevoli lavoratori, non si capisce per quale motivo vi è una equiparazione sul piano sanzionatorio quanto meno delle sanzioni accessorie pesanti e significative all'ipotesi non commendevole dal punto di vista giuridico; ciò è tanto vero che esiste nella legislazione attuale e viene confermato in questo disegno di legge un intervento sanzionatorio. Ma per quale motivo vengono equiparate due ipotesi di reato assolutamente incomparabili, una meno grave e una più grave? Non vi è alcuna giustificazione. Non solo. Il rischio concreto di altrettante concrete ingiustizie Nel decreto flussi integrativo per il 2006 è stata realizzata per via amministrativa una serie di incongruenze operative che ha portato a non aver ancora esaurito il numero di domande, da parte dei datori di lavoro, di impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri. Ci sono liste d'attesa e file da oltre un anno, derivanti non dalle norme del Testo unico sull'immigrazione, ma dall'incapacità di gestire la loro applicazione. Ricordo che cinque anni fa, per la regolarizzazione degli extracomunitari, un numero un numero molto più significativo di lavoratori stranieri da regolarizzare e di incombenze qualitativamente più rilevanti fu esaurito in un tempo certamente inferiore. Ora immaginiamo un datore di lavoro, anche domestico (per usare la terminologia impropria della lettera *a*) del primo comma di questo articolo), che, spinto dalla necessità, impieghi alle proprie dipendenze attraverso l'illecita intermediazione - e magari non coglie neanche il carattere di illiceità di questa intermediazione - un lavoratore straniero e si vede applicare tutte le sanzioni accessorie, che sono davvero pesanti e sono state immaginate originariamente per un reato - questo sì - veramente grave e odioso quale il grave sfruttamento di lavoratori stranieri. Tutto ciò rende assolutamente inammissibile anche un lontano consenso a questa norma, che non può che andare incontro ad una sonora bocciatura. È l'unico esito che merita.

poc'anzi rilevato in relazione ad una diversa considerazione del lavoro svolto tra le mura domestiche rispetto a quello svolto in un'impresa industriale o commerciale, ai fini della sanzione per il datore di lavoro. Ove anche si considerasse in modo diverso un'*enclave* familiare rispetto ad un'attività imprenditoriale, è comunque eccessiva la sanzione, che viene fissata, con emendamento del relatore, da 3000 a 5000 euro; è eccessiva perché introduce in una fattispecie semplice una discrezionalità che non ha ragione di essere ed è eccessiva perché, con riferimento all'attività

un'ora al giorno per le pulizie di casa e una badante per eventuale ausilio notturno) introduce una fattispecie di portata enorme sotto il profilo pecuniario, ferma restando la diversa considerazione del lavoro svolto tra le mura domestiche rispetto a quello svolto in un'impresa commerciale o industriale sotto il profilo dello sfruttamento. C'è di più: al comma 3, lettera *d)*, che introduce l'articolo 2-*bis*, c'è una esenzione dalla sospensione delle attività, cioè della sanzione interddittiva, per le imprese agricole che svolgono attività con ciclo biologico e allevamento del bestiame.

Ci si rende conto che sono proprio quelle le imprese dove il caporalato opera di più? *(Commenti dai banchi del Gruppo Ulivo).* Ci si rende conto che in Campania, Sicilia e Calabria sono imprese che utilizzano il caporalato di tipo mafioso quelle di allevamento del bestiame, quelle di ciclo biologico, visto che ci sono gli aiuti europei verso cui tutte queste imprese si indirizzano? Ci si rende conto che le si fa continuare a lavorare? Allora, mi chiedo perché

nel mercato del lavoro italiano una quantità enorme di persone, spesso irregolari, invece, si vuole assolutamente restringere la normativa sull'impiego delle stesse e - io aggiungo - giustamente se la prima fase del fenomeno

perché deve esserci differenza nel trattamento di chi impiega irregolarmente un cittadino extracomunitario e di chi fa lo stesso con un cittadino italiano. italiano. Facciamo qualcosa di gravemente lesivo nei confronti di quei cittadini italiani appartenenti alle fasce più deboli, i giovani senza ancora una occupazione stabile, i cinquantenni espulsi dal mercato del lavoro, che si trovano esattamente nella stessa situazione. Qualche mese fa fece scalpore - poi, ovviamente, non se ne fece più nulla la notizia riportata dai giornali che tra i dipendenti diretti, cioè i cosiddetti collaboratori o portaborse dei parlamentari, 600 erano senza contratto. Poiché il centro-destra non ha 600 parlamentari, vuol dire che una bella fetta di questi sono o erano collaboratori di parlamentari di centro-sinistra. Non capisco, allora, perché i parlamentari di centro-sinistra propongano e votino una legge che mette in galera un imprenditore che assume

si trova di fronte ad un provvedimento di sequestro. L'impresa continua a produrre. Il criminale mafioso, quindi, che ha realizzato ed organizzato quell'impresa con crimini efferati, che possono andare dal sequestro di persona alla rapina, dal traffico di droga al traffico di armi e anche di esseri umani, esseri umani, in realtà vede, mediante questa legge, previsti per la sua attività criminale, e la collaterale attività imprenditoriale, provvedimenti sanzionatori molto, ma molto meno pesanti di quelli stabiliti, invece, per un imprenditore che ha avuto l'avventura, la sventura, l'imprudenza - possiamo anche la marcia convenienza - di assumere uno, due, tre lavoratori extracomunitari, illegalmente soggiornanti, reclutati da un caporale che, appunto, è oggetto e perseguibile di denuncia penale. Mi chiedo come sia possibile che in questo il Paese un'impresa che derivi la sua attività dai profitti criminali sia meno sanzionabile di un'impresa che impegna

vera ragione di questo disegno di legge, ma in questi termini, rispondendo a questi interrogativi, allora può darsi che il mio voto di astensione potrà anche trasformarsi in un voto di sostegno. Presidente, anch'io intervengo per annunciare il mio voto di astensione, in quanto questo disegno di legge, in particolare l'articolo 2, va in direzione opposta a quello che dovrebbe essere lo spirito della legge.

volontariato porterà a un'azione che sarà comunque illegale, maggiormente illegale, e che tenterà di superare queste norme,

Presidente, dovrei fare un appello ad alcuni colleghi che hanno tirato in ballo la mia povera nonna. Caro Mantovano, caro Galli, vi chiedo, per cortesia, di lasciare in pace queste povere vecchiette. C'è già tutto il centro-sinistra che le tiene affamate e le mette in croce,

Bene hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto a ricordare come, in particolare per quanto riguarda le fasce più deboli, legate non soltanto ai livelli reddituali ma anche all'età, si si giunga di fatto a una sostanziale equiparazione anche in termini sanzionatori con lo stesso datore di lavoro. Voglio altresì se non emerge in modo evidente, una chiara ed identica disparità di trattamento tra il lavoratore straniero e il cittadino italiano, l'applicazione di sanzioni che arrivano al limite del grottesco: basterebbe infatti rendersi conto che un'applicazione fiscale del comma 12-*ter* potrebbe portare addirittura, in una lettura concatenata dei vari commi, al sequestro preventivo di un'abitazione;

viceversa, stanno cercando semplicemente di sopravvivere, niente di più, signor Presidente. Un provvedimento deve avere una sua *ratio*, una sua logica, deve produrre effetti precisi. Questo testo non farà altro che aggravare situazioni di illegalità; andrà ingiustificatamente a colpire fasce più deboli e a creare discriminazioni tra il cittadino italiano e il lavoratore straniero. Allora, se il principio di per sé in astratto può essere condivisibile, non ne è certamente condivisibile l'impalcatura e questo spiega e motiva il mio voto di astensione.

applicarlo in termini rigorosi, tuttavia non comprendo una cosa. Lei sta concedendo a tutti i senatori che intervengono in dissenso il tempo di tre minuti.

e non è questo il caso di specie, perché non vi è né limitazione né esclusione - «un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di dieci minuti».

un potere discrezionale di aumento del tempo a disposizione del parlamentare per effettuare il suo intervento, ma non di restrizione del tempo stesso. L'ultima parte dell'articolo 109, comma 2, testualmente afferma: «Uguale facoltà» - cioè quella di intervenire per dieci minuti - «è riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte Presidente, se il mio intervento può essere considerato ostruzionistico, ma non conoscendo la prassi del Senato, mi chiedo: a fronte di una disposizione così chiara del Regolamento, che nel conferire al Presidente un potere discrezionale di aumento del tempo a disposizione del singolo intervenuto, come mai ella ritiene invece di dover restringere questo tempo da dieci a tre minuti, 2, del Regolamento del Senato che il senatore che interviene in dissenso, quando non vi è contingentamento dei tempi, ha gli stessi diritti del senatore che interviene a nome del Gruppo? Aggiungo, signor

il parlamentare, in ossequio al dettato costituzionale che lo fa rispondere solo alla Nazione, scioglie - sia pure temporaneamente - il nodo con la disciplina del partito perché attraverso quel suo intervento, per l'appunto, si dissocia dalla linea ufficiale del Gruppo. Le chiedo quindi, Presidente, se vi sono precedenti o meno, se vi è un articolo diverso che sostenga la sua decisione e mi scuso per averle fatto perdere del tempo. Senatore Palma, la ringrazio molto del suo intervento, che è oltremodo opportuno, anche perché mi da l'opportunità di chiarire, forse ad altri colleghi dell'Aula che stanno partecipando ai nostri lavori, come stiamo procedendo. Ho seguito esattamente questo criterio e questo principio: innanzitutto, mi sono avvalso di una norma consuetudinaria, se così si può dire, relativa al fatto che tutte le dichiarazioni in dissenso molto normalmente avvengono con un consenso degli stessi dichiaranti il loro voto di dissenso, con l'attribuzione di un tempo per queste dichiarazioni che in genere è di uno, due, tre, al massimo cinque minuti; è una norma consuetudinaria. Mi sono avvalso di questa facoltà che è stata tacitamente accolta da tutti i colleghi. Mi sono soprattutto avvalso, però, di un'altra norma nel Regolamento, che lei ha tralasciato nel suo intervento, anche se sono certo che non

di armonizzare i tempi della discussione sulla base del calendario concordato e definito, in questo caso unanimemente dalla Conferenza dei Capigruppo.

il Regolamento, cercando di armonizzare i tempi degli interventi, per rispettare i termini del calendario. Non so se riusciremo in

far perdere del tempo al nostro Senato che però oggi affronta un tema quanto mai delicato. Vorrei ricordare a tutti noi, e a me per prima, l'articolo 17 della legge finanziaria, che è stato approvato da quest'Assemblea

delle donne immigrate, avvalendosi di un nuovo strumento messo in atto dalla finanziaria, e che, recuperando risorse dalle liquidazioni dei *supermanager*, poteva utilizzare tali fondi a favore della formazione, anche professionale, delle donne immigrate regolarmente presenti nel nostro Paese.

dovremmo e potremmo aiutare nel modo più efficace. La modalità prevista da questo provvedimento rischi a invece di vanificare uno sforzo che tutti stiamo compiendo, nel tentativo di amalgamare quelle politiche del lavoro previste per i cittadini italiani e le cittadine italiane con quanto invece in materia di lavoro deve poter riguardare anche gli ospiti del nostro Paese, spesso preziosi al nostro sistema economico e industriale, in particolare nel settore dei servizi. Ho l'impressione che questa legge non si ponga, invece, il problema di cogliere il vero risultato: tanti più immigrati potranno lavorare regolarmente, tanto migliore sarà la qualità del nostro mercato del lavoro. Con questi articoli vessatori e a senso unico otterremmo lo stesso risultato che abbiamo ottenuto rispetto alla situazione delle donne italiane nel mondo del lavoro, che infatti rappresentano la più bassa percentuale d'Europa,

Signor Presidente, ho colto una nota di rammarico in codesta Presidenza nel momento in cui, visto l'intervento sul Regolamento svolto dal senatore Palma, il mio intervento era stato dato per fatto ed ella ha consentito l'intervento della senatrice Bonfrisco. Mi onora il fatto che l'intervento della senatrice Bonfrisco, non soltanto come augusta collega ma anche per la qualità dell'intervento, probabilmente è stato di maggiore interesse rispetto al mio che cade, come quello della settimana precedente, alla chiusura della seduta, laddove la lancetta più lunga si sta lentamente ma inesorabilmente posando sulla cifra più alta del quadrante. Ringrazio il vice

in quanto facente parte della Commissione affari costituzionali, probabilmente si attesta in una posizione di difesa della dichiarazione di voto fatta dal nostro Gruppo in quella Commissione. ella, però, ha detto che probabilmente, chiamato ad impegni ancor più importanti in Commissione antimafia o altrove, non ha perfetto ricordo di quello che è avvenuto. Io invece so che in quella sede alcuni colleghi, non volendosi proporre all'opinione pubblica come contrari ad una persecuzione ancora più incisiva nei confronti del caporalato, si sono astenuti. Quel che, però, non soddisfa la mia attenzione e la mia curiosità è che questa maggioranza soltanto nell'intervento del professor Treu ci ha dato un qualche chiarimento di come si è formato l'articolato che stiamo esaminando; un articolato per quanto

Presidente, vorrei forzare la sua cortesia, perché d'altronde non è che riusciamo ad esitare il provvedimento non ha più motivo di esserci, perché quale armonizzazione del calendario, se abbiamo finito di discutere del provvedimento? Non c'è nessuna votazione, quindi dibattiamo di quello di cui non abbiamo dibattuto, nel senso che abbiamo parlato soltanto noi: ma il dibattimento significa dialettica ed abbiamo osservato che, a parte l'intervento del professor Treu, nessuna ricerca della permanenza sul contrario è stata fatta in quest'Aula. La nostra è una posizione soltanto unilaterale, continuiamo a chiedere che il Governo ci ripensi e a dire che il provvedimento è fatto male, ma la maggioranza e il Governo non ci danno chiarimenti in proposito. Allora, signor Presidente,

La Presidenza del Senato non ha nessuna difficoltà a cercare di sapere come sono andate le cose e a riferirgliele